Comunico che, in data 24 luglio 2021, è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»

Signor Presidente, il testo del decreto-legge, all'esito delle numerose integrazioni effettuate dalla Camera, si compone di 121 articoli. Si tratta di un numero di articoli pari a 54 in più rispetto ai 67 della versione originaria del decreto-legge nel complesso i commi aggiuntivi ammontano a 177, mentre originariamente erano 215. Il testo, che, come si vede, è particolarmente esteso e complesso, è stato trasmesso al Senato, come anche lei ha ricordato, sabato 24 luglio e il termine per la conversione scadrà fra tre giorni, venerdì 30 luglio: pertanto, pena la sua decadenza, dovrà essere approvato dal Senato in brevissimo tempo, senza ulteriori modifiche. La prassi ormai invalsa di concentrare l'esame di merito dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge in una sola Camera, su cui si potrebbero aprire articolate riflessioni, in questo caso non ha e non avrebbe consentito di completare la trattazione in Commissione, pur senza apportare modificazioni. Il provvedimento è stato incardinato nella seduta odierna della Commissione; è stata svolta la discussione generale, ma non è possibile procedere oltre con l'esame. una nuova finestra"). Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Parrini, il disegno di legge n. 2332, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Comincini. Ne ha facoltà.

aiutarci ad imprimere e determinare una svolta nella costruzione del futuro del nostro Paese, perché, se è vero che nel corso di questi mesi ci siamo sempre ripetuti quanto fosse importante essere riusciti a portare a casa ingenti risorse dalle istituzioni europee, è altrettanto vero che, per scaricare sui territori i miliardi del *recovery plan*, c'è bisogno di regole chiare e di una macchina amministrativa capace di fare fronte alle sfide che ci attendono. Da questo punto di vista, l'articolo 1 del decreto fornisce, al primo comma, le finalità del decreto-legge, volto a definire il quadro normativo nazionale per semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti, nell'ordine: il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Piano nazionale per gli investimenti complementari e il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030. In quest'Aula in molti abbiamo avuto la fortuna di vivere un'esperienza da sindaco o da amministratore locale e sappiamo bene quante difficoltà ci siano nel rapporto tra investimenti, pubblici o privati che siano, pubblica amministrazione e cittadini, le quali nel corso degli anni si sono tradotte in ritardi cronici, che hanno dunque spesso significato inefficienza e mancato sviluppo. In Italia, in media, per le grandi opere pubbliche i tempi di approvazione sono arrivati a raggiungere i sedici anni, un tempo inutilmente e infinitamente lungo per un Paese che vuole avere l'ambizione di ripensare il proprio futuro e che deve farsi trovare pronto alla grande sfida della transizione ecologica e digitale e della messa in sicurezza dei nostri edifici, ma che deve anche risolvere l'atavico problema della sicurezza ambientale. Su questo punto specifico, la seconda parte del decreto, che riguarda le semplificazioni le semplificazioni ordinamentali legate alla transizione ecologica e alle procedure di modifica del codice dell'ambiente, nella parte relativa alle norme concernenti le opere pubbliche per l'attuazione del PNRR, ci dà risposte importanti. Allo stesso tempo, penso anche, nello specifico, al grande tema del dissesto idrogeologico, che pure è stato toccato in questo provvedimento grazie al lavoro dei colleghi del Partito Democratico nell'altro ramo del Parlamento. Siamo tuttavia consapevoli, e ce ne siamo accorti ogni volta che abbiamo provato a fare interventi di questo tipo, di quanto sia difficile tenere in equilibrio l'esigenza di velocizzare, semplificare, sburocratizzare il più possibile le procedure amministrative e, allo stesso tempo, garantire la piena tutela dei lavoratori e soprattutto il pieno rispetto della legalità. È un provvedimento, quello che stiamo discutendo, sul quale, come sempre più spesso accade, non abbiamo avuto la possibilità di intervenire. Nonostante alla Camera sia stato fatto un gran lavoro di implementazione rispetto al testo varato dal Governo e di grande mediazione fra le forze politiche rispetto a temi specifici che, a mio avviso, hanno migliorato il provvedimento stesso, resta il problema, sempre più acuto, di un monocameralismo alternato perfetto.

che aver previsto una *governance* partecipata, non solo dal Parlamento, ma anche da tutte le forze del Paese, rappresenti una garanzia per tutti i cittadini. Parimenti, mi sembra rilevante avere previsto che la gestione dei fondi e di tutti i processi collegati abbia il Parlamento come protagonista in tutte le sue tappe. Il provvedimento in discussione prevede che il Governo sia chiamato a fornire alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sul PNRR, per migliorarne le criticità e per svolgere un ruolo sinergico con entrambi i rami del Parlamento. che sia una previsione di assoluta importanza, anche rispettosa delle funzioni che ci vengono attribuite dalla Costituzione. Sappiamo bene che, quando il Parlamento viene messo nelle condizioni di svolgere bene il proprio compito, il Paese ne beneficia anche in termini di trasparenza, essendo Camera e Senato i luoghi deputati, i luoghi simbolo della discussione e del confronto. Ritengo poi degno di nota il risultato che si è conseguito anche grazie al lavoro del collega Ceccanti alla Camera e che, all'articolo 8-*bis*, si traduce nell'introduzione di un obbligo, in capo al Governo, di trasmissione al Parlamento di relazioni periodiche, che ci facciano comprendere meglio a che punto siamo con la produzione dei provvedimenti attuativi, che, come sappiamo tutti molto bene, tanto spesso sono l'ostacolo ultimo alla realizzazione di moltissime iniziative, che, pure se deliberate dal Parlamento, restano ferme al palo. Passando invece agli articoli che compongono il capo VII del provvedimento in esame, ovvero le disposizioni in materia di efficienza energetica, vediamo che queste ultime sono in larga parte destinate ad accompagnare alcuni interventi specificamente elencati nel PNRR. Tra questi, come accennavo all'inizio del mio intervento, troviamo quelli legati alla transizione energetica e alla mobilità sostenibile. Su questi temi saremo chiamati, sempre più frequentemente, a scelte non semplici, ma di assoluta rilevanza. L'ultimo G20 sull'ambiente, gli accordi sul clima e il piano Fit for 55 tracciano il solco dei confini entro i quali saremo chiamati a fare le nostre scelte. Appare chiaro che costruire un sistema più semplice, con un apparato burocratico meno lento e macchinoso, significa anche essere in grado di raggiungere, prima e meglio, quegli obiettivi che, in ambito europeo e internazionale, l'Italia si sta impegnando a raggiungere. Penso, ad esempio, a tutto il tema legato alla decarbonizzazione e all'utilizzo delle fonti rinnovabili. Altrettanto importante è la previsione di cui all'articolo 33, che riconosce la detrazione al 110 per cento (il cosiddetto superbonus), anche per gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente a quelli antisismici. Essa si accompagna anche all'ulteriore semplificazione della disciplina per fruire del superbonus, stabilendo che, attraverso una comunicazione di inizio lavori asseverata, la CILA, è possibile attestare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, rendendo così non più necessaria l'attestazione dello stato legittimo. Di pari rilevanza appaiono gli articoli seguenti del provvedimento, che mirano a semplificare e a disciplinare meglio aspetti rilevanti legati alla gestione dei rifiuti. Penso dunque all'articolo 34, sulla *end of waste*, oppure ancora al dissesto idrogeologico e allo sblocco delle grandi opere e delle infrastrutture, per le quali il provvedimento in esame prevede procedure speciali, fino ad arrivare alle modifiche per i contratti pubblici, cioè quelle al codice degli appalti su cui, come sappiamo, sappiamo, c'è un impegno del Governo. Su tali modifiche mi pare vi sia stato un giudizio positivo anche da parte dell'ANCI, che si è vista accogliere diverse proposte miranti a semplificare il lavoro di migliaia di sindaci, i quali, ancora di più in questa fase, saranno chiamati a svolgere un ruolo di prim'ordine. Nel corso di questi mesi, la nostra Assemblea ha visto l'approvazione di provvedimenti indubbiamente rilevanti. Ritengo che quello che stiamo discutendo oggi possa tranquillamente essere annoverato tra questi ultimi. il nostro Paese ha un ritardo imperdonabile, che, quando si trasforma in inefficienza, determina la rottura di quel patto di fiducia che si instaura tra lo Stato e i cittadini e che va preservato, mostrando efficienza e serietà, perché è proprio in questa rottura che poi si inseriscono le organizzazioni criminali e che si alimenta la corruzione. Credo di poter dire che con questo provvedimento contribuiamo a tenere saldo quel patto tra Stato e cittadini, con l'ambizione di immaginare e costruire nel migliore dei modi il futuro delle generazioni che verranno.

il secondo decreto-legge semplificazioni che transita in questa legislatura. L'esame del primo era stato di stretta competenza del Senato, mentre questo della Camera devo dire che Forza Italia ha provato in tutte e due le occasioni a inserire quella che abbiamo sempre ritenuto la semplificazione regina e in assoluto principale,

Sono state accolte altre indicazioni, per noi fondamentali, sulla questione del superbonus al 110

con le decine di migliaia di persone che ci lavorano? Non siamo contenti di questo, ma siamo convinti che l'impegno che abbiamo richiesto potrà vedere la luce nel prosieguo. Ci preoccupa un po' la questione del subappalto.

che non possono necessariamente competere con i grandi *general contractor* che hanno tantissimi avvocati e commercialisti, ma zero operai. Questo è un problema e lo segnaliamo in maniera costruttiva, perché non va assolutamente bene mettere le piccole imprese nelle condizioni di essere strangolate dai grossi gruppi, che prenderanno gli appalti e poi faranno il subappalto fino al 100

Dobbiamo avere procedure semplificate, come accade in tutto il mondo: avendo un occhio anche all'estero per le mie attività, vi dico francamente che per realizzare un edificio, aprire un'attività o consentire la partenza di un'impresa non servono due anni e mezzo di carte, ma bastano due giorni e mezzo. Questo accade perché ci sono regole chiare, quindi apri e poi vengono a controllarti con calma (addirittura, ti chiedono l'appuntamento per venire a verificare se l'aspetto sanitario funziona). Siamo contenti. La semplificazione va nella giusta direzione, ma c'è una cosa che ci preoccupa ulteriormente: tutto finirà nel 2026. Non va bene. Forza Italia farà una battaglia perché la semplificazione sia moltiplicata, vada nella direzione della continuità e consenta alle imprese di avere veramente una prospettiva che garantirà occupazione, lavoro, sviluppo e certamente un'economia forte. Abbiamo due alternative: o cala il debito (impossibile) o aumenta il PIL. Noi siamo per la seconda opzione.

le cose semplici sono quelle più difficili da farsi; quindi, quando si intraprende quella per la semplificazione, è sempre una strada difficile. Tuttavia, adesso è assolutamente necessario, perché

servono strumenti che consentano una snellezza operativa che non può essere quella che abbiamo vissuto nei decenni scorsi. Colleghi, prima

per gestire i lavori pubblici. È chiaro che strumenti del genere non sono più adeguati, quindi con il decreto-legge al nostro esame ci apprestiamo a superare queste difficoltà.

un tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale; un'unità di *audit* che svolgerà attività di controllo sull'attuazione del PNRR, un'unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e l'ufficio per la semplificazione. Ci sarà anche un ufficio di monitoraggio e rendicontazione, che dovrà tenere conto dei vari stati di avanzamento, perché è all'Europa che dovremo rispondere dell'avanzamento delle spese. In quest'ambito, viene anche istituita una soprintendenza speciale e ci saranno alcuni strumenti - rispetto ai tempi previsti, stiamo andando parecchio avanti - perché, per il superamento di eventuali dinieghi o dissensi da parte di organi dello Stato, il Presidente del Consiglio dovrà intervenire entro cinque giorni, tempi ai quali sicuramente in passato non siamo stati abituati.

energetica e anche alla promozione dell'energia circolare, attraverso una più efficiente gestione e il riutilizzo dei rifiuti. Ci saranno anche interventi e misure per la diffusione delle comunicazioni digitali nella pubblica amministrazione. Oggi, nonostante l'evoluzione del digitale, abbiamo ancora uffici che spesso non comunicano fra loro. Ecco che allora questa rappresenta una misura assolutamente utile. un processo di snellimento nelle procedure di gara anche per importi più piccoli, quindi per favorire le piccole aziende e imprese italiane.

sui lavori che possono essere concessi in subappalto, purché l'amministrazione committente stabilisca quali sono le opere che non possono essere subappaltate.

cento, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per le ONLUS. Auspico che questa cabina di regia, il segretariato tecnico e i vari organi costituiti riescano a comunicare in maniera costruttiva fra loro e che queste misure vengano prorogate vengano prorogate oltre i termini necessari allo sviluppo e all'attuazione del PNRR.

Signor Presidente, colleghi, il ruolo della Lega al Governo è di responsabilità e controllo per il bene dell'Italia. Ripartire con il Covid-19 che ancora incombe sulle nostre vite e avere comunque un fiume di risorse del Piano non lascia il tempo per opportunità politiche, a prescindere. Il nostro compito primario è solo quello di collaborare per migliorare provvedimenti che rimarranno regole per la crescita e soprattutto debiti economici e culturali per i nostri figli. Ammettiamo sia necessario, perciò, convertire in legge con urgenza il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, ovvero il decreto semplificazioni-*bis*, perché reca disposizioni opportune anche per la gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nel provvedimento si definiscono i rapporti tra le amministrazioni e il monitoraggio e il dialogo con le autorità europee, lasciando la cabina di regia a vari Ministri e Sottosegretari guidati dal Presidente del Consiglio. di oltre 200 miliardi di euro: circa 65 di sovvenzioni e 130 di prestiti; circa un miliardo e mezzo di *just transition fund* e 13,5 di React-EU. Sono un fiume di soldi, strutturato e semplificato in sei missioni. Se però nella vita pubblica e amministrativa non siamo pronti e preparati, questo fiume si seccherà, lasciandoci privi di strutture e vantaggi e solo con debiti, problemi e rimpianti. semplificazioni-*bis*, infatti, continua nello snellimento delle procedure burocratiche. Vediamo di buon'occhio, tra le novità presenti nei 67 articoli

Quest'ultima lascia così spazio a migliori interventi di efficientamento energetico e sismico, perché sono da sempre complessi e onerosi: si valutano in circa 110 milioni, che possono così essere messi a disposizione per le migliorie. la massima semplificazione per gli investimenti in edilizia libera, per i quali basterà una semplice descrizione e dichiarazione. Si conferma il superbonus per l'eliminazione delle barriere architettoniche, che si estende inoltre, per attività di prestazioni di servizio sociosanitari e assistenziali e per immobili quali - ad esempio - collegi, convitti, orfanotrofi, ospizi, caserme, conventi, case di cura e ospedali per gli addetti ai lavori nelle categorie B1, B2 e D4. L'ampliamento della semplificazione riguarda anche la digitalizzazione: dall'articolo 38 sulle notifiche digitale agli atti della pubblica amministrazione. Vi sarà l'introduzione della possibilità di delegare, a mezzo DSG (sistema di gestione deleghe) ad altro soggetto, l'accesso per il proprio conto o servizio *on line* e di conferire, modificare o eleggere il proprio domicilio digitale. Nell'articolo 38-*ter* è previsto, per i gestori di servizio di pubblica utilità e agli operatori di telefonia di reti televisive e comunicazioni, l'obbligo di trasmettere agli utenti in tempi opportuni (almeno quaranta giorni) l'eventuale sospensione delle forniture. Gli articoli 38 e 39 39 sono propedeutici se vogliamo veramente autostrade digitali per la pubblica amministrazione. Si riduce a tre mesi, partendo da sei mesi, il termine per la conclusione dei procedimenti in materia di installazione di reti di comunicazione elettronica.

Seneca diceva che non è vero che abbiamo poco tempo: la verità è che ne perdiamo molto. Ed allora svegliamo gli anestetizzati del reddito di cittadinanza e iniziamo a lavorare tutti, perché c'è molto da fare. *(Applausi)*. PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà. Presidente, membri del Governo, colleghi, vorrei concentrare il mio intervento sul tema dei lavori pubblici e provare a interpretare la visione del MoVimento 5 Stelle sulle fasi di realizzazione di un'opera da parte della pubblica amministrazione. lavori pubblici nel decreto-legge semplificazioni rivestono un ruolo di primaria importanza. L'enorme quantità di denaro che stiamo per ricevere dalla Comunità europea non va semplicemente speso, ma deve essere per l'Italia una forma di investimento che dia immediate ricadute sull'economia del Paese per un immediato rilancio. Per questo le semplificazioni possono essere intese non come una mera spinta alla spesa rapida e forsennata, ma come una vera e propria proiezione al futuro di quello che sarà il patrimonio infrastrutturale del Paese. Per avere un'infrastruttura resiliente e che garantisca longevità bisogna necessariamente partire dalla centralità della progettazione, perché un progetto concepito e fatto perbene permetterà di avere un'infrastruttura rispondente alle finalità per le quali è stata ideata. La centralità del progetto è quindi un vero e proprio dogma, e la vera necessità sarebbe quella di revisionare il codice degli appalti. Sarebbe essenziale avere essenziale avere tre codici diversi e distinti rispetto a quello attuale, che invece racchiude in sé lavori, servizi e forniture. Ognuno di questi tre settori ha una specificità e peculiarità diversa ed è per questo motivo che andrebbero distinti nettamente tra loro. Per quanto riguarda il subappalto, in questo decreto-legge se ne modifica la disciplina con alcune norme che entrano in vigore immediatamente ed altre che hanno efficacia differita, a decorrere dal 1° novembre 2021. vi è la norma che dispone che, fino al 31 ottobre 2021, il subappalto passerà dal 30 per cento ad un massimo del 50

possiamo accettarlo, anche se per il MoVimento 5 Stelle l'ideale sarebbe stato restare alle soglie già valutate e ponderate in precedenza: quindi non uno zero per cento, ma neanche un 100 per cento, come chiede l'Europa. L'ideale sarebbe stato proprio restare come già definito e, quindi, su una quota del 30 o 40 per cento in ordinario. Perché mi soffermo su questo? È molto semplice. Noi vogliamo evitare che le società di finanza facciano letteralmente impresa, stravolgendo le regole del mercato. E ciò perché in Italia abbiamo la fortuna di avere un artigianato delle costruzioni di altissimo livello, un artigianato industriale quasi manifatturiero. E l'aumento delle soglie del subappalto va a sfavore di queste realtà; va a svantaggiare chi realmente realizza un'opera imprese che invece è giusto remunerare bene e che non devono vedere limati i loro compensi per effetto del meccanismo del subappalto, che tutto favorisce, fuorché esse, Per quanto riguarda il tema dell'appalto integrato, ovvero mettere a gara un progetto che non è esecutivo, in questo decreto si prevede di andare in gara per le opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Fondo complementare

la stazione appaltante valuterà i progetti definitivi e le offerte e incaricherà l'impresa non solo del lavoro, ma anche del progetto esecutivo, liquidando il progetto definitivo già presentato. La seconda possibilità, invece, è quella che la stazione appaltante inviti le imprese a fare un'offerta senza nemmeno fare un progetto definitivo e questo per il MoVimento 5 Stelle è assolutamente da evitare, in quanto viene meno il concetto espresso in precedenza di centralità della progettazione. Ci auguriamo comunque che le stazioni appaltanti facciano esclusivamente ricorso alla prima opzione, lasciando la seconda solo in caso di straordinaria emergenza. Infine, c'è il tema della trasparenza, che è di rilievo assoluto. decreto sblocca cantieri abbiamo introdotto il concetto di offerta più congrua, norma che peraltro sta portando ottimi risultati, dati alla mano. Il metodo dell'offerta più congrua non ha alcuna difficoltà di applicazione; basta utilizzare una formula molto semplice, che taglia automaticamente le ali, escludendo le offerte anomale e in una sola giornata permette di individuare l'aggiudicatario dell'appalto tra le imprese che hanno partecipato al bando. Con il metodo dell'offerta più congrua di fatto si aggiudica la gara con un ribasso più prossimo al ribasso medio e non al massimo ribasso. Basta, quindi, con il massimo ribasso, che ha ridotto il settore degli appalti ad una giungla. Presidente, nell'esprimere rammarico per le modalità con cui non ci viene permesso di lavorare in questo ramo del Parlamento su un decreto così importante per la gestione dei fondi del PNRR e per il Fondo complementare al PNRR, devo riconoscere che, rispetto al testo base, molto è stato migliorato, anche se non tutto. Un ulteriore vaglio da parte di questa Camera avrebbe rafforzato la qualità e l'effetto dell'ennesimo decreto semplificazioni. Detto ciò, come Commissione lavori pubblici, lo spettro del massimo ribasso lo abbiamo lasciato nelle bozze che circolavano nei giorni che hanno preceduto il varo del decreto da parte del Consiglio dei ministri. Mi auguro, quindi, che questa dinamica, molto simile a quella di un monocameralismo, venga al più presto superata.

Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, il senatore Mallegni ha detto che è la seconda volta che affrontiamo il tema della semplificazione. Ha ragione, però, questo decreto è molto più di un testo sulla semplificazione: è un atto obbligatorio, dovuto per dare attuazione ai progetti del *recovery plan* e per tirare i primi 25 miliardi degli oltre 200 dei fondi europei. Fuori dai tecnicismi, perché sarebbe abbastanza complicato e non c'è il tempo, e dalle critiche che si possono sicuramente muovere, perché zone d'ombre ci sono -una di queste è sicuramente il tema del subappalto, sul quale personalmente non la penso come senatore Mallegni, nel senso che la corresponsabilità tra appaltatore e subappaltatore nei confronti del committente merita di essere attenzionata, chiaramente con un intervento sulla rete della filiera - mi concentrerò su tre atteggiamenti che - secondo me - il Governo ha tenuto per mettere in evidenza il valore del decreto in questione: un atteggiamento consapevole e sincero, un atteggiamento di collaborazione

vorrebbero investire, è proprio la qualità dell'attività legislativa che va assolutamente migliorata, e - secondo me - anche attraverso azioni di *benchmark* internazionale. Apro una piccola parentesi sul codice degli appalti: pensate che in Germania conta solo 100 articoli e da noi ne conta 200, per cui gli spazi per migliorare sarebbero tanti. Altra osservazione: i canali straordinari, quali l'istituzione della cabina di regia, i comitati interministeriali, i gruppi di controllo e di monitoraggio, i poteri autocertificativi del silenzio-assenso riconosciuti ai privati sono sicuramente, di nuovo, la consapevolezza di dover dare una risposta pragmatica e concreta a un sistema che fatica a essere snello, flessibile, veloce ed

se non vengono nel frattempo progressivamente semplificate, potrebbero far nascere il rischio che l'Italia nel 2026, anziché essere estremamente veloce,

aspetto è la collaborazione: con il tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale che ha funzioni consultive nelle materie collegate all'attuazione del *recovery plan* si riconosce specificatamente il valore della collaborazione, che personalmente considero estremamente positiva, tra pubblico e privato, tra mondo politico e mondo scientifico, tra imprese e lavoratori, tra società civile e Governo. Ora, se questa collaborazione mette in evidenza, con riferimento alle parti in causa, gli aspetti migliori delle parti considerate, e quindi pone ai margini rivalità e antagonismi che non servono assolutamente a nulla e non sono proficui alla creazione di un modello virtuoso, secondo me la strada è proprio quella giusta. Vi è infine l'aspetto del pragmatismo che è stato introdotto in maniera scientifica nei contratti pubblici, che vengono intesi non

che hanno al loro interno una serie di parametri dei quali non possiamo assolutamente fare a meno, perché denotano il mondo moderno e contemporaneo. Mi riferisco alle politiche di assunzione che privilegiano i giovani, la parità di genere, la conciliazione della vita privata con il lavoro.

la pubblica amministrazione su un binario non straordinario, ma ordinario di velocità, secondo me questo Paese può ritornare a crescere e quel debito di cui siamo tutti consapevoli potrà effettivamente essere ripagato grazie alla crescita del PIL.

mia e del mio Gruppo per questo Piano nazionale con il quale sono stati predisposti numerosi progetti per il nostro Paese per l'attuazione del *recovery fund*, approvato poco più di un anno fa,

Con questo risultato abbiamo tutelato la dignità del Paese e l'autonomia delle istituzioni comunitarie. Il Governo italiano è forte e l'approvazione di questo Piano ne rafforza l'azione. Ora, per noi, c'è la responsabilità di far ripartire al meglio l'Italia. «Dobbiamo correre»:

grazie al quale l'Italia potrà vivere una stagione di riscatto economico mediante - finalmente - investimenti europei che devono trovare una loro piena ed efficiente attuazione. Se il presidente Conte ha ottenuto una capacità di spesa di notevole rilievo mai vista prima, il presidente Draghi e l'attuale Governo hanno varato un Piano nazionale denso di investimenti che, nel corso degli anni, potrà ridurre il *gap* economico accumulato rispetto agli altri Paesi europei e aggravato dalla devastante pandemia. Dico anche: ricordiamoci il Sud Italia. Entrando nel merito del decreto-legge in vorrei soffermarmi sulle misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure che questo Governo ha introdotto. Tra i tanti strumenti previsti, di dirimente importanza è sicuramente l'ampliamento dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione pubblica. Non ne possiamo più della burocrazia. L'espressione «potere sostitutivo» ricomprende istituti diversi afferenti ai rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni e privati. Quanto alla natura giuridica, si tratta, pur nella sua varietà, di un potere inquadrabile nell'ambito dei controlli. Ecco, dunque, individuata la *ratio* principale di questo strumento: vigilare affinché le risorse ottenute dal *recovery fund* siano spese in maniera celere ed efficiente. Tale potere, inoltre, si articola in modo diverso, assumendo caratteristiche specifiche e ulteriori a seconda dell'ambito di applicazione. L'elemento comune è rappresentato dalla sostituzione di un soggetto a un altro nello svolgimento di una determinata attività in conseguenza della mancata adozione, con rapidità ed efficienza, nei termini previsti di atti rientranti nella competenza di un'altra amministrazione, ovvero nell'adozione di atti non conformi al paradigma normativo. Il decreto-legge disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato in caso di inadempienza di un soggetto attuatore di progetti o interventi del PNRR, ovvero qualora sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali dello stesso. La norma specifica che l'inadempienza può concretizzarsi in presenza di mancato rispetto di un obbligo assunto; mancata adozione di atti prodromici all'avvio di progetti; inerzia e ritardi nell'esecuzione dei progetti. In ogni caso, condizione per esercitare il potere sostitutivo è che sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano. In tali casi, il Presidente del Consiglio, su proposta della cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Questo principio andrebbe applicato a tutti i procedimenti amministrativi del nostro Stato. Nel caso in cui il soggetto attuatore continui a non provvedere, il Consiglio dei ministri individua il soggetto cui attribuire, in via sostitutiva, il potere di provvedere ad adottare gli atti o i provvedimenti necessari o all'esecuzione dei progetti. L'individuazione del soggetto a cui affidare il potere sostitutivo avviene sentito il soggetto attuatore. Questi soggetti possono essere un'amministrazione, un ente o un organo, un ufficio, ovvero uno o più commissari *ad acta* appositamente nominati. Dunque, si tratta di una misura importante, volta a semplificare e accelerare l'attuazione del PNRR. In relazione a siffatto potere sostitutivo di natura amministrativa, si possono distinguere vari ambiti di applicazione, i quali vengono ricostruiti alla luce della particolare articolazione dei rapporti di diritto pubblico che possono venire in rilievo. Nei rapporti orizzontali tra amministrazioni, ai fini dell'adozione di decisioni pluristrutturate, viene di rilievo il silenzio-assenso tra amministrazioni *ex* articolo 17-*bis* della legge n. 241 del 1990. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti in esame, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. Si tratta di un potere sostitutivo la cui funzione è semplificare il procedimento decisionale consentendo l'adozione dell'atto finale. Nei rapporti tra amministrazione e privati vengono in rilievo i termini per la conclusione del procedimento. Se l'amministrazione competente non conclude il procedimento entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge n. 241, è previsto l'intervento sostitutivo di altro soggetto inserito nell'ambito della stessa struttura organizzativa. Se vengono in rilievo procedimenti rilevanza economica di cui all'articolo 4 della legge n. 124 del 2015 e al regolamento n. 194 del 2016, è previsto l'intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha natura giuridica di alta amministrazione. Le modifiche introdotte, dunque, determinano conseguenze rilevanti sui poteri sostitutivi enunciati, attuabili in caso di inerzia dell'amministrazione a provvedere. Con un'unica modifica il Governo ha previsto che il potere sostitutivo possa essere attribuito non solo a una figura apicale, ma anche a un'unità organizzativa. In secondo luogo, si introduce la possibilità che l'attuazione del potere sostitutivo possa avvenire anche d'ufficio, oltre che su istanza del privato. Questa mia breve esposizione sulla natura del potere sostitutivo, sul suo concreto operare, sulle novità introdotte da questo decreto testimoniano che la centralità dell'amministrazione pubblica nell'attuazione del Piano nazionale è fondamentale. Il Governo ha voluto dunque ampliare la portata del potere sostitutivo mediante modifiche che, inserendosi nei procedimenti amministrativi in generale, garantiscono celerità, efficacia ed efficienza nell'attuazione dei progetti contenuti nel Piano nazionale. Non disperdiamo ciò che il presidente Conte ha fatto per l'Italia. Signor Presidente, nell'illustrazione che ha fatto il relatore c'è la dimensione di quanto ci fosse da semplificare e peraltro quanto ancora ci sia. ricordato quanti articoli siano stati aggiunti nel passaggio parlamentare. Che poi questo sia avvenuto alla Camera piuttosto che al Senato poco importa alla società, agli operatori, alle aziende, ai Comuni. Spesso queste sono cose del fatto che siano giuste - appassionano noi, ma molto di meno la società e chi subisce le scelte legislative del Parlamento. È stato detto che il motivo - non voglio dire il pretesto - è quello del PNRR,

abbiamo appena scalfito la situazione. Mi fa piacere che la collega del MoVimento 5 Stelle abbia finalmente preso coscienza che c'è la necessità di mettere mano al codice degli appalti. Forse si è persa qualche decina di interventi della Lega in questi tre anni *(Applausi)*, oppure qualche riunione di maggioranza, quando stavamo insieme al Governo. Se siamo in ritardo di tre anni, è perché quando la Lega, con forza, ha posto sul tavolo la necessità di rivedere perché no? Per una volta va detto - in ottica europea il problema del codice degli appalti, non è stato fatto. Basterebbe stracciare quello che c'è, che non semplifica e ritarda e nemmeno dà garanzie sul piano della lotta alla corruzione e al malaffare, e prendere le linee generali che valgono in Europa. Non è mai troppo tardi, si potrebbe cominciare a farlo ora. Del resto - magari questo è sfuggito ai più, perché è notizia di appena una settimana fa

mostruosa di 109 miliardi a carico delle aziende; praticamente, metà del PNRR potremmo darlo indirettamente alle aziende semplicemente non pesando negativamente, come purtroppo lo Stato sta facendo. Peraltro, è in quel tessuto che che trovano spazio la corruzione e il malaffare; è in quel tessuto che le piccole e medie imprese, i piccoli e medi Comuni, quelli che hanno più difficoltà, non riescono a difendersi da quelle realtà che sanno dove infilarsi. Per questo sarebbe importante fare ancora di più sulla semplificazione, a cominciare dal codice degli appalti.

sancito il criterio, il principio per cui si parte dalle opere che hanno maggiore incidenza sul piano economico e maggior ritorno per il Paese; è esattamente il contrario di quello che avviene oggi, perché fino a oggi tanto più grande è l'opera, tanto più è divisiva, tanto più si rinvia e si manda la palla a bordo campo. Sarebbe facile citare il treno alta velocità (TAV) o il ponte sullo Stretto di Messina. Finalmente si stabilisce un criterio.

fatto sul dissesto idrogeologico, ma meglio di me lo dirà il collega Pazzaglini che ha seguito per noi questo tema. Ci sono, dunque, degli spunti positivi anche se si poteva fare di più. Del resto, questo è un Governo di coalizione. Non è tutto quello che noi avremmo voluto, ma sicuramente non rinunciamo a tante delle proposte che la Lega ha fatto e che speriamo possano trovare spazio in altri provvedimenti. Peraltro, per fare qualcosa di rivoluzionario in Italia ci sarebbe non da produrre altre leggi, ma da tagliarne centinaia, migliaia (peraltro in quest'Aula c'è chi

il Parlamento approva una legge di delegazione europea. Ebbene, forse bisognerebbe approvare tutti gli anni una legge di semplificazione che, di volta in volta, possa sistemare la legislazione vigente. Questo sì che semplificherebbe la vita di cittadini, famiglie e imprese e non è mai troppo tardi per cominciare a farlo.

l'obiettivo enunciato dal decreto-legge in esame è assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Di certo, è un obiettivo condivisibile per fare questo, si sono allargate di molto le maglie: io faccio riferimento ai settori di mia competenza e penso - per esempio - che alcuni pareri del Ministero della cultura non saranno più considerati vincolanti (articolo 30); sono stati ridotti i tempi procedimentali riguardanti la verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 44); si prevedono casi in cui i poteri delle sovrintendenze possano essere avocati o sostituiti da una nuova sovrintendenza speciale.

Faccio mia la riflessione del presidente Mattarella quando, nell'ultima lettera indirizzata ai Presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi, ribadisce che la necessità di attuare speditamente il programma di investimenti e riforme concordato in sede europea non può affievolire il dovere al rispetto della Costituzione. Dunque, per quanto riguarda i settori di mia competenza, io richiamo assolutamente l'articolo 9, che chiede a noi parlamentari e al Governo di rispettare il nostro patrimonio e garantire la tutela del nostro patrimonio artistico e del paesaggio, ma anche l'articolo 32, che ci impone di tutelare la salute. la salute. Sullo sfondo del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli obiettivi di questo decreto-legge, c'è un obiettivo primario, che è la lotta globale ai gas climalteranti. Ciò significa combattere il surriscaldamento globale e cercare di contrastare così i fenomeni climatici estremi e avversi dovuti ai cambiamenti climatici. Dunque, dobbiamo fare molta attenzione, perché questo chiaramente ci impone un efficientamento energetico. Ma dobbiamo anche fare attenzione che la nostra necessità di decarbonizzare e di efficientare la produzione energetica da fonti di energia rinnovabili non possa, in qualche modo, andare a compromettere la biodiversità, gli ecosistemi - di cui l'Italia, tra l'altro, vanta il primato in Europa per numero - e l'ambiente in generale. Vi porto un esempio. Pensate a 90 ettari di foresta, che producono annualmente circa tra le 10 e le 20 tonnellate di ossigeno e assorbono annualmente circa tra le 5 e le 10 tonnellate di CO2. Pensate se quei 90 ettari, che in totale assorbirebbero 657 tonnellate di CO2 e ne rilascerebbero 450 di ossigeno, fossero compromessi e rasi al suolo per fare un impianto industriale eolico, con un impiego di 600 metri cubi di cemento per ogni plinto delle 8 pale eoliche e, dunque, anche con un rischio per le conseguenze di sussistenza e sopravvivenza degli ecosistemi e della biodiversità. Questo potrebbe accadere sul crinale del Mugello, per esempio. esempio. Colleghi, dobbiamo fare molta attenzione. Qui siamo tutti d'accordo sulla necessità di semplificare e sulla necessità di una transizione ecologica, ma questa non può che avvenire nel rispetto della biodiversità, degli ecosistemi, degli ambienti e delle attività, anche microeconomiche, che sussistono in quegli *habitat* e in quegli ambienti. Altrimenti, se noi pensiamo di realizzare la transizione ecologica senza porci il problema dell'impatto sull'ambiente e sulle comunità, ci troveremo di fronte, anzi immersi fino alla punta dei capelli in un grande paradosso ecologico

Signor Presidente, signora rappresentante del Governo, colleghi e colleghe, voglio fare due ragionamenti, uno di metodo e uno di merito. Lo abbiamo già ripetuto più volte in quest'Aula, ma purtroppo siamo stati unica *vox in deserto clamantis* e non credo che le cose Ci troviamo a dover discutere - più che altro a prendere atto - della conversione di un decreto-legge senza che questo ramo del Parlamento possa muovere una foglia; possa intervenire con un minimo di emendamento; possa rendere compatibile un provvedimento di questo genere con le necessità che la storia di ognuno di noi, in quest'Aula, ha maturato. Molti di noi sono stati amministratori comunali, provinciali e regionali e quindi sanno perfettamente, a proposito di sburocratizzare e snellire le procedure, quali sono le esigenze e le aspettative. Il provvedimento in esame necessitava di un robusto intervento parlamentare, e cioè dei rappresentanti dei cittadini, perché molte volte i provvedimenti sono figli della burocrazia ministeriale, soprattutto quando i capi dei Ministeri sono non politici, ma persone della società civile e quindi ostaggio - se mi è consentito il termine - dei burocrati dei loro Ministeri. Ecco allora che la funzione del Parlamento è proprio attualizzare e trasferire quella mole di esperienza, che ognuno di noi ha maturato nella sua attività politica, nei provvedimenti che servono ai cittadini. Quindi, mi auguro di non essere più costretti a esaminare provvedimenti a scatola chiusa, con tutto il rispetto del lavoro fatto dai colleghi della Camera dei deputati, che hanno quasi raddoppiato il numero degli articoli. Questa è la questione di metodo. la questione di merito, non possiamo che essere favorevoli a un intervento che mira non soltanto a velocizzare

sia esso imprenditore, utente o persona qualunque, non è più visto come colui che vuole frodare lo Stato, il Comune o l'amministrazione: è visto come una persona con la quale si deve collaborare. Quindi, è la pubblica amministrazione ad essere al servizio del cittadino e non viceversa. Probabilmente c'è voluta l'autorevolezza del presidente Draghi, ma c'è voluta anche la spada di Damocle

a scadenza, ai 209 miliardi di euro. Allora ben venga questa situazione: può darsi che non tutti i mali vengano per nuocere, se il nostro Paese cambia e inverte la rotta. Ci sono molte iniziative nel provvedimento in esame che sono stati cavalli di battaglia del nostro Gruppo, del nostro movimento, del nostro partito, a partire appunto dai tempi certi nel rilascio di autorizzazioni e nella valorizzazione del silenzio-assenso della pubblica amministrazione. È chiaro che il Governo si è dovuto munire di una serie di organismi che hanno il compito di controllare e verificare in concreto l'andamento dell'esecuzione e della realizzazione dei progetti, che sono sempre conseguenza della necessità di ottenere quelle somme. Anche a tale proposito, ci siamo sempre riempiti la bocca transizione ecologica e del cambio di marcia rispetto all'essere schiavi dell'energia fossile, ma abbiamo creato una serie di paletti per le energie rinnovabili. Tutti vogliamo liberarci dalla schiavitù del carbone, ma nessuno vuole realizzare sul proprio territorio i parchi eolici o i pannelli fotovoltaici. Pertanto, questo intervento

abbiamo bisogno di fare passi avanti molto importanti, e mi auguro che queste norme non abbiano la vita

Ne cito una fondamentale. È stata stabilita la norma per la quale non è possibile fare ricorso al TAR e avere la sospensiva per un'opera che riguarda il PNRR. Ebbene, tutte le attività della pubblica amministrazione, perché questo è veramente un cancro che impedisce lo sviluppo del nostro territorio. Quindi, mi auguro che le misure previste siano l'inizio di una nuova stagione

dà attenzione al nostro Paese, all'Italia tutta, quindi anche al Mezzogiorno. In modo particolare, il testo dedica alcuni articoli al Mezzogiorno laddove considera la riforma, sebbene come inizio, delle ZES, delle aree interne,

Che cosa voglio dire in quest'Aula, Presidente? In realtà il problema per il Mezzogiorno è stato rappresentato da due figure: da un lato, i pontificatori pessimisti; dall'altro, i governanti incapaci. Chi sono i pontificatori pessimisti? Quelli che devono creare per forza il *pathos*, senza il quale la sceneggiata non viene fuori per bene, bene, e che dicono sempre che c'è qualcosa che non va; si sforzano di mettere in campo filosofie molto articolate, in alcuni casi anche distorte, ma mai azioni concrete in grado di garantire crescita e sviluppo. Per esempio, i pontificatori pessimisti attuali sono coloro i quali vorrebbero fare cartastraccia della riforma del procedimento penale della Cartabia; cosa che non sta né in cielo né in terra perché è una riforma importante per il nostro Paese, ma anche e soprattutto per il PNRR. Poi ci sono i governanti incapaci, quelli che hanno avuto in questi anni milioni e milioni di

condotta idrica per portare acqua nei campi - ci vogliono venti-trent'anni, qualcosa evidentemente non ha funzionato. Mettiamo i puntini sulle "i" rispetto all'emendamento di cui parlavo prima. Un emendamento sottoscritto anche dalla Lega, che inserisce all'interno dell'articolo 2, il comma 6*-bis*, che provo a segnare in stampatello cosicché i terroristi psicologici che stanno all'esterno possano capirlo,

comprendere che questa è un'occasione storica per l'Italia, ma ancor di più per il Mezzogiorno. È un'occasione storica per accorciare le distanze tra i territori, che non si può consumare come è stato fatto in passato. Noi siamo ancora nell'obiettivo 1. Ricordo che quando la mia Regione tornò nell'obiettivo 1 vi fu un'esultanza generale da parte di quella classe dirigente di sinistra che amministrava la nostra Regione; esultava, perché non percepiva che

da poter spendere, più o meno alla bisogna, senza una visione strategica. Questo è il punto di demarcazione, oltre il quale non si può più andare adesso. Ora o mai più. Ora o mai più. Visione, coraggio e responsabilità. *(Applausi)*. Qual è la ricetta? Basta con il piagnisteo stucchevole di questi pontificatori tristi e pessimisti. Basta con l'incompetenza cronica di governanti incapaci, che sono aridi nelle idee e immobili nell'azione. Andiamo avanti con i costruttori di futuro, perché hanno orgoglio e fierezza. Questo è quel che serve all'Italia; questo è quel che serve al Sud.

di fondi che arriveranno al nostro Paese grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza, avuti - ricordiamocelo sempre - grazie all'eccellente lavoro svolto dal precedente Governo Conte II, sostenuto dal MoVimento

alle sanatorie e ai condoni edilizi. Non è così. Dobbiamo dirlo subito e lanciare il messaggio giusto. Il superbonus del 110 per cento non intacca in alcun modo le sanatorie e i condoni. Per questo motivo devo intervenire, per ristabilire una sorta di operazione verità. Ricordo che già nel settembre 2018, con il decreto-legge Genova, alcuni gridarono

il decreto-legge semplificazioni-*bis* non c'è alcun tipo di sanatoria, non c'è alcun tipo di condono edilizio. Ma soprattutto ribadiamo che, fin quando il MoVimento 5 Stelle farà parte di un Governo di questo Paese, queste cose non le vedremo mai.

Immaginiamo che oggi, sebbene siamo in un periodo di scia della crisi economica e pandemica (perché ancora non è stata superata), oltre 4 miliardi di euro riconosciuti come cessione del credito di imposta. Sapete perché sono soltanto quattro? Perché il Governo ancora non assicura la proroga della scadenza del superbonus almeno al 2023. Basta pensare che oggi il settore delle costruzioni è così determinante al punto da segnare un più 36 per cento su base annuale: sono numeri enormi. Avevamo già ascoltato le voci di chi ci chiedeva aiuto per semplificare le procedure sul superbonus e una proposta concreta l'avevamo già fatta nel decreto-legge sostegni con un emendamento del MoVimento 5 Stelle, che proponeva che per gli interventi su cui riconoscere il superbonus bastasse una semplice comunicazione di inizio lavori asseverata, perché erano paragonati a interventi di ristrutturazione edilizia. È molto semplice: si tratta di manutenzione straordinaria, un po' come quando qualcuno di noi deve fare il rifacimento dell'intonaco a casa o deve sostituire le tegole sul manto di copertura. Quella è una manutenzione straordinaria che si fa con la cosiddetta CILA. In più abbiamo non è richiesto lo stato legittimo dell'immobile. Questo non significa che si può fare su un immobile illegittimo; non è richiesto lo stato legittimo dell'immobile e alle colleghe che ridono chiedo di leggere bene l'articolato. Bisogna solo Bisogna solo attestare il titolo abilitativo, l'autorizzazione dell'ultimo provvedimento o se la casa è stata realizzata prima del 1° settembre 1967.

e magari in qualche unità abitativa qualcuno non vuole far entrare il tecnico perché ha l'altezza difforme internamente da quella che ha comunicato al Comune o che qualcun altro ha le verande abusive (il principale abuso in Italia forse avviene sulle verande). Perché Giuseppe e tutto il condominio su tutta la parte comune legittima non deve vedersi riconosciuto il superbonus 110 per cento? Non c'è motivo. Tutti noi siamo stati bombardati da *e-mail* che richiedevano aiuto in questo senso

Il superbonus non intacca dunque né la legittimità dell'immobile, né l'illegittimità dell'immobile, né parti illegittime dell'immobile stesso. Questo sia chiaro.

parlamentari, si prevede la possibilità di intervenire anche su eventuali irregolarità emerse dai controlli *ex post*. Le violazioni formali non inficiano tutto il superbonus, ma gravano solo sulla irregolarità riscontrata, ed in caso di violazioni decade il beneficio solo sulla parte parte contestata e non sul complesso dell'agevolazione. È facile, semplice ed elementare, e chi fa finta di non vedere gioca sporco. Con un emendamento consentiamo di andare in deroga alle distanze nel caso di realizzazione del cordolo antisismico o del cappotto termico, come diamo la possibilità fino a trenta mesi di cambiare la residenza per chi compra una casa su cui si si opera con il superbonus. Le imprese anche di ristrutturazioni immobiliari che abbattono e ricostruiscono possono avere trenta mesi di tempo se usufruiscono del superbonus. Infine, vi sono alcune informazioni sull'edilizia libera, che è valida purché nella CILA

a eliminare nella valutazione della fattibilità dell'opera le piccole difformità, che già non erano considerate. Di Ischia parleremo in un altro momento.

Nella relazione illustrativa della 1a Commissione, si dice molto chiaramente, nero su bianco, che la prassi ormai è che sia solo una Camera a valutare i provvedimenti. Questo è gravissimo, perché stiamo mettendo in atto delle riforme costituzionali di fatto, se abbiamo visto che il popolo italiano si era espresso diversamente, ma il tempo è poco. questo provvedimento tende a semplificare l'*iter*, perché è necessario realizzare le opere e investire investire i soldi che ci vengono dal PNRR nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi. È giustissimo, chi potrebbe non essere d'accordo su questo? Lo sottoscrivo, metodo è assolutamente sbagliato. Innanzitutto è un metodo vecchio e quindi anche verificato, non è solo errato per una valutazione che ci viene da un pregiudizio. Esso

nascono proprio nel 1991, quando Guido Carli scriveva a «la Repubblica» una lettera su come vi fosse necessità di una crescita zero del numero dei dipendenti pubblici e di privatizzare, di colpire le pensioni e i salari e, ancora, di contenere di contenere le retribuzioni entro il tasso programmato di inflazione. Nel prossimo triennio tra cessazione di servizio, collocamento e riposo dovremmo avere 200.000 dipendenti in meno. Come potevamo credere che la pubblica amministrazione - le

bisogna sostituire quella parte politica che da due decenni tende a dare spazio al *welfare* in parole povere, perché bisogna scoraggiare la tendenza ad avere

realizzato alcuno degli obiettivi che si poneva. Infatti, Cantone la dichiarò criminogena e venne abrogata, anche se con il decreto-legge sblocca Italia si cercò di mantenere molte di quelle semplificazioni. Cosa faceva la legge obiettivo? Comprimeva la partecipazione pubblica, comprimeva la valutazione ambientale e azzerava la pianificazione urbanistica.

dimostrato il loro fallimento, anche perché, nel momento in cui non c'è la partecipazione pubblica, sappiamo per certo

significativo. Questo è fondamentale, perché tutta l'espletazione di questo programma va esattamente nella direzione di arrecare un danno significativo: per il consumo del suolo, per la sanatoria di alcune opere abusive e sicuramente, anche per quanto riguarda la transizione energetica, va

già segnalato dall'Europa come un PNIEC da rimodernare e da riguardare secondo i nuovi obiettivi che si è data l'Europa. all'Europa per i nuovi obiettivi, però il PNIEC si troverà sicuramente ad affrontare

si era riusciti a far uscire dal PNRR la cattura della CO2, bocciata dall'Europa e dalla

Avremo bonifiche parziali, senza valutazione del rischio, che verranno quindi estrapolate dal totale. C'è la possibilità di bruciare il CSS in impianti non autorizzati, ossia senza la necessità di una revisione sostanziale. Non ho dubbi che questa scelta ci porterà fuori strada: sia dalla strada dell'accelerazione sui tempi e dell'efficientamento delle realizzazioni, ma anche fuori strada per quanto riguarda tutti gli obiettivi ambientali. Questo è veramente molto grave.

la nostra cultura enogastronomica e le nostre tradizioni, si pensa purtroppo anche alla nostra burocrazia. Impossibile nasconderlo: la nostra è una burocrazia da *record*. Bisogna prenderne atto, fare *mea culpa* e procedere con azioni necessarie per cambiare lo stato dei fatti, come ci chiedono cittadini e imprese. Faccio parte di un Gruppo parlamentare - Forza Italia - che non si è mai astenuto dal far notare determinati *bug* di sistema e ha sempre lavorato per fornire soluzioni concrete, ora più che mai con i nostri Ministri e Sottosegretari, che stanno svolgendo un lavoro egregio. È il caso di quanto fatto dal ministro Brunetta, fin dal primo giorno all'opera per cercare di rendere efficiente il funzionamento della pubblica amministrazione. Il decreto-legge oggi in esame è frutto del suo lavoro, di concerto con gli altri Dicasteri, a cui estendo la mia gratitudine del sottosegretario Bergamini, presente in quest'Aula. Credo che il segreto per il buon funzionamento di quest'esperienza di governo sia custodito in una frase pronunciata dal presidente Draghi:

in quelle parole sono custoditi i sogni delle giovani donne e giovani uomini, dei nostri imprenditori e lavoratori. In questo senso, nazionale di ripresa e resilienza costituisce un unico volano da sfruttare appieno e non sono ammessi errori. Lo scorso marzo, durante gli Stati generali del Sud, ho avuto modo di confrontarmi con gli attori coinvolti nel sistema di mobilità, i quali hanno espresso le preoccupazioni comuni a tutti. Unanime era la richiesta di snellimento delle procedure e svecchiamento legislativo, perché con le procedure in vigore oggi le opere infrastrutturali con un costo superiore a 100 milioni di euro hanno un tempo di realizzazione medio di circa sedici anni.

qualche numero in modo da essere più chiara. La burocrazia costa alle imprese italiane 57 miliardi di euro l'anno e questo è un vero e proprio limite alla piena espressione del nostro potenziale economico. A causa della troppa burocrazia, dalla quale derivano inefficienze e scarsa qualità, l'Italia perde ogni anno 70 miliardi di euro È quindi evidente che un intervento volto a limitare questi sprechi sia ora più che mai essenziale, alla luce dello sforzo economico che si richiederà alle future generazioni. esame, rendendo possibile l'anticipo di 25 miliardi di euro dei fondi europei in arrivo, è la garanzia che l'Italia dovrà procedere in velocità, senza pregiudicare le legittime tutele per le imprese. Il cambio di passo è evidente: dimezzati i tempi delle valutazioni ambientali, semplificate le procedure autorizzative che riguardano anche la produzione di energia da fonti rinnovabili e ridotte le attese per le autorizzazioni per la banda ultralarga. Si accelerano gli appalti e le realizzazioni di importanti opere strategiche per l'intero Paese, semplificando, tra l'altro, le procedure per le opere di impatto rilevante (penso, ad esempio, all'alta velocità sulla tratta Salerno-Reggio Calabria). il Governo ha mantenuto la promessa di sbloccare il superbonus del 110 per cento, che è un importante incentivo per l'efficientamento energetico e gli interventi antisismici sugli edifici. Riguardo agli interventi antisismici, in particolare relativi agli edifici pubblici, faccio una richiesta all'Esecutivo. Qualche mese fa si è concluso il quadriennio del finanziamento per gli interventi di adeguamento antisismico degli edifici scolastici diverse sono le amministrazioni che, a causa degli evidenti rallentamenti degli *iter* burocratici causati anche dalla situazione emergenziale ancora in atto, sono decaduti dal finanziamento. Chiedo quindi ai rappresentanti del Governo qui presenti uno sforzo al fine di superare questa difficoltà burocratica e consentire di utilizzare il denaro stanziato fino all'ultimo centesimo. Così facendo, consentiremo ai nostri figli, a partire dal prossimo anno accademico, di studiare in luoghi più sicuri. Naturalmente è tutto da considerarsi come un primo importante passo in direzione della complessa semplificazione della macchina burocratica che attendiamo ormai da troppo tempo. A questo - ne sono certa - seguiranno altri concreti e incisivi provvedimenti per far ripartire il nostro Paese in una carreggiata senza deviazioni o inversioni di marcia. La corsa dell'Italia non dovrà più arrestarsi.

dai gravi eventi meteo e non solo, al popolo sardo che da giorni sta lottando contro incendi distruttivi, alle comunità flagellate da piogge torrenziali e tempeste che hanno determinato esondazioni, frane e crolli, con pesanti danni.

il nuovo decreto semplificazioni, peraltro senza aprire i termini neanche per gli ordini del giorno in Commissione, unici residuali spazi di manovra che erano rimasti a noi senatori. Purtroppo il ruolo di ratificatori di Palazzo Madama proseguirà la prossima settimana con il decreto che istituisce l'Agenzia sulla cybersicurezza. Comunque sia, semplificazioni dell'era Draghi è un provvedimento corposo e significativo, che dimostrerà molta più efficacia del decreto semplificazioni dello scorso anno, varato dall'Esecutivo Conte-*bis* che, annunciato in pompa magna, ha poi deluso le aspettative. Il decreto contiene molte norme importanti che introducono la Commissione VIA per i progetti PNRR-PNIEC, con il *fast track* dei procedimenti prioritari, nuove semplificazioni per il super bonus, nuove semplificazioni per gli impianti rinnovabili, nuove semplificazioni per l'economia circolare, per l'economia montana e forestale, per interventi di manutenzione e sistemazione idraulica in aree montane ad alto rischio idrogeologico. Importante anche la norma riguardante lo sviluppo del sistema energetico della Sardegna *(Applausi)*, con la previsione dell'emanazione di un molti sono consapevoli che per il *phase out* del carbone sull'isola e per avere garanzie per lo sviluppo industriale del Sulcis e non solo, il gas naturale dovrà giocare un ruolo importante. Il decreto semplificazioni è funzionale a mettere a terra gli obiettivi del PNRR, in particolare quelli della missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», che con 70 miliardi è tra le sei missioni quella più significativa. Il decreto è funzionale anche per attuare il Piano nazionale integrato energia e clima, che è in corso di revisione per effetto dei nuovi *target* europei, il taglio a meno 55 per cento di CO2 al 2030. Gli obiettivi di efficientamento energetico e rinnovabili, già sfidanti, saranno rivisti - e di molto - al rialzo. Da notare, però, che mentre si semplifica la Regione Lazio amministrata dal MoVimento 5 Stelle e dal Partito Democratico, partiti che più di altri spingono sulle rinnovabili, decide in questi giorni una moratoria di un anno per autorizzare impianti fotovoltaici. *(Applausi)*. Evidentemente, siamo già ai primi cortocircuiti. Le parole d'ordine di questi tempi sono ormai sostenibilità, transizione ecologica, decarbonizzazione per contrastare i cambiamenti climatici. Sono parole risuonate nello scorso *week-end* anche al G20 di Napoli, le cui conclusioni però hanno evidenziato l'esistenza di profondi distinguo, anzi divergenze con le posizioni assunte e confermate da Cina, India e Russia. Partendo da qui, occorre seriamente riflettere se puntare ciecamente agli obiettivi di decarbonizzazione che Bruxelles si è data, senza considerare quello che fanno gli altri *player* globali. In questa fase caratterizzata dall'emergenza sanitaria, che ha determinato una profonda crisi economica, occorrono crescita e occupazione. Con la svolta *green*, occorre evitare bagni di sangue, con l'affossamento di nostre filiere. Occorre dunque, per una transizione sana ed ecologica, adottare pragmatismo, bandendo l'ideologia ambientalista, spesso anti-impresa. *(Applausi)*. Occorre pensare a *policy* che coniugano sostenibilità ambientale, economica e sociale; applicare il principio della neutralità tecnologica e soprattutto, nel portare avanti la transizione ecologica, occorre fare attenzione ad un lato oscuro e ai più sconosciuto della stessa: il monopolio cinese. I veicoli elettrici, gli impianti fotovoltaici e i parchi eolici richiedono molti più minerali rispetto alle controparti basate sui combustibili fossili. Rispetto a un'auto convenzionale, un'auto elettrica richiede sei volte gli *input* di minerali; rispetto ad un impianto a gas, un impianto fotovoltaico richiede sette volte più risorse minerali, un impianto eolico *on-shore* nove volte e addirittura 15 per l'eolico *off-shore.* Queste non sono affermazioni della Lega, lo si legge nel recente rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia. Il passaggio a quello che molti dipingono come un sistema energetico pulito determina un significativo fabbisogno di rame, litio, nichel, cobalto, zinco e terre rare. inevitabile, dunque, che la richiesta crescente di queste materie prime, vero e proprio monopolio della Cina, che possiede anche molte concessioni minerarie in Africa, determinerà lo spostamento del baricentro della geopolitica mondiale. dovremo certamente realizzare *gigafactory* per produrre batterie, pannelli fotovoltaici, elettrolizzatori per idrogeno, ma comunque sia ci legheremo mani e piedi al gigante d'Oriente per metalli e minerali. Occorre saperlo.

rischia di aumentare le già forti asimmetrie esistenti nel mondo globalizzato. Portare avanti a tappe forzate il *green deal* europeo senza che le altre potenze economiche facciano lo stesso, come purtroppo il recente G20 dimostra, espone l'Europa ad un forte rischio di catastrofe economica, senza che l'ambiente ne benefici in alcun modo, perché il nostro sforzo verrà vanificato. Per Pechino, seconda economia mondiale e primo produttore di anidride carbonica (con il 28 per cento), oggi la priorità non è decarbonizzare, ma costruire ancora centrali a carbone per produrre energia elettrica a basso costo, perché l'energia elettrica è un importante fattore di produzione. Per questo in un simile contesto internazionale, in assenza di garanzie e impegni precisi e condivisi da parte di tutti, l'Europa deve essere prudente nel cercare di essere la prima della classe, perché le *policy* troppo spinte verso la decarbonizzazione stanno determinando forti aumenti di prezzo delle quote di

ma ad ottobre, con l'ultimo quadrimestre, che cosa succederà? La corsa al rialzo dei prezzi dell'energia non si fermerà e questo metterà ulteriormente in ginocchio le nostre imprese, già fiaccate dalla emergenza Covid. L'Europa, che di fronte a questi enormi rischi dovrebbe dunque puntare ad una transizione ecologica graduale e condivisa, purtroppo è pervasa da un'ideologia ambientalista, come dimostrato dalla recente proposta della Commissione europea con il pacchetto Fit for 55. scheme* (ETS) ad altri settori porterà ulteriori rincari per tutti, mentre la previsione della messa al bando dal 2035 delle auto a combustione interna è pericolosa e inaccettabile. Abbandonare auto a benzina, a gasolio, a GPL, a metano, anche quelle ibride di ultima generazione, in favore solo di quelle elettriche, molto costose e fuori dalla portata della maggior parte dei cittadini, significa fermare gli investimenti in ricerca e sviluppo, uccidere la nostra filiera dell'*automotive* e soprattutto quella della raffinazione, che si sta riconvertendo alla produzione di carburanti *low carbon.* Occorre sfatare il mito delle auto a spina ad emissione zero ed imporre il *life cycle assessment* per la valutazione del ciclo di vita e degli impatti emissivi del processo che porta produzione, esercizio, manutenzione e demolizione di un prodotto, cioè la macchina a batteria elettrica. *(Applausi)*. Si scoprirebbe allora che anche un'auto elettrica inquina, e non e non solo perché è alimentata ad energia elettrica prodotta in gran parte da fonti fossili. Il Governo italiano agisca, dunque, in sede europea per arginare questi *diktat.* La decarbonizzazione deve essere portata avanti con pragmatismo, applicando il principio della neutralità tecnologica, sapendo che non è possibile elettrificare tutto, a partire dai settori energivori *hard to abate,* come la siderurgia, la chimica, il cemento, il vetro, la carta e la ceramica, per i quali nella lunga attesa dello sviluppo dell'idrogeno a costi competitivi, il ruolo del gas naturale sarà strategico, almeno fino al 2050.

per semplificare la normativa, il Governo ha varato un provvedimento, che si è arricchito di ulteriori norme nel passaggio alla Camera, e arriva quindi ricco di ben 222 pagine di

Nel frattempo, però, tutti gli uffici pubblici, gli uffici dei Comuni, i privati e le aziende dovranno studiare 222 pagine

di questo ormai sistematico monocameralismo di fatto, il Senato è totalmente esautorato. Per questo, i componenti della maggioranza si troveranno a dover votare norme che neppure loro hanno avuto il tempo di leggere, tantomeno di analizzare, né, comunque, di modificare;

Nel frattempo, però, l'aggravio per i cittadini è notevole. La lettera inviata dal Presidente della Repubblica ai Presidenti di Senato e Camera in questi giorni,

Questo decreto-legge dovrebbe recare misure di *governance* (naturalmente, perché in italiano, a quanto pare, non esiste la parola governo o governanza) del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Ebbene, nonostante questo titolo molto ampio, sarebbe lungo l'elenco degli articoli e dei commi che non hanno nulla a che fare con queste indicazioni. Qual è il problema? Il problema è che la Costituzione e la giurisprudenza Corte costituzionale dicono che bisogna fare altrimenti e anche la lettera del Capo dello Stato dice che bisogna fare altrimenti. Il problema è che non ci sono garanzie per i cittadini. Non vi è garanzia che le norme siano fatte con un certo criterio, che siano leggibili con un minimo di di facilità e con un approccio minimo al quale non sia necessario affiancare una serie di ricerche, che oggi, grazie a Internet, si fanno velocemente, ma non sempre. Tra queste misure, poi, vengono introdotte, anche modifiche pressoché costituzionali, perché la cabina di regia presidenzialista che viene delineata non è una cosa da poco, visto che gestisce le enormi risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il fatto è che,

è, se tutto resta in capo al Governo e se il Parlamento è lì solo per dire sì a scatola chiusa, si pone un problema di tenuta istituzionale. Per fare un esempio di ciò che può essere infilato in un provvedimento, quando si schiaffano 222 pagine di norme, tutte in un colpo solo, sotto un titolo generico, cito l'articolo 47-*ter¸* cheho visto

e, di conseguenza, essendo all'opposizione, Fratelli d'Italia voterà ovviamente contro. Del resto, a scatola chiusa non compriamo nulla e se poi, quando apriamo la scatola, vediamo cose di questo tipo, allora siamo veramente e fermamente convinti, sempre di più, della nostra posizione all'opposizione.

e individua misure di semplificazione delle procedure amministrative, necessarie all'attuazione di un piano ambizioso. Si tratta di purtroppo, come ormai spesso accade, in Senato è meramente formale, in una sorta di dimensione nuova, che viviamo - quella di un monocameralismo di fatto - ma che è comunque fondamentale, per dare il via ad un provvedimento che permette al nostro Paese di farsi trovare pronto per la sfida del PNRR, a cui molto abbiamo lavorato nei mesi scorsi, anche in sede parlamentare, per definire programmi, misure

di regia presso la Presidenza del Consiglio, che dovrà consentire una centralizzazione delle funzioni di indirizzo nei confronti dei vari soggetti che saranno chiamati a dare attuazione al Piano e che dovrà fungere anche da stanza di compensazione delle eventuali criticità che dovessero insorgere, e che pure sono in qualche modo immaginabili. Bene anche la valorizzazione del ruolo delle Regioni, dei Comuni, delle Province e dei soggetti del partenariato economico, sociale e territoriale, anch'essi chiamati a dare il loro contributo nella cabina di regia. Bene anche il titolo II della parte prima sui poteri sostitutivi che specifica un un punto che avevamo segnalato nelle nostre relazioni in fase di predisposizione del PNRR. Si prevede infatti che, qualora la mancata azione di Regioni o enti locali in qualità di soggetti attuatori metta a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali, operi una procedura di sostituzione dell'amministrazione inadempiente affinché, anche tramite un commissario *ad acta*, siano adottati gli atti necessari all'esecuzione dei progetti. Come tutti i colleghi e le colleghe sanno, sono stati due i punti che che abbiamo e che ho cercato in prima persona di valorizzare in questi mesi. Il primo è il rilancio del nostro Mezzogiorno. Non mi stancherò di parlare di questo. Molto è stato detto e scritto sul fatto che il PNRR rappresenti un'occasione unica per avviare il rilancio del Mezzogiorno e per la ripresa del processo di convergenza con le aree più sviluppate del Paese. Lo abbiamo rappresentato con forza nei documenti parlamentari e in tutte le iniziative politiche che abbiamo portato avanti in questi mesi. Anche oggi, nella Commissione che mi onoro di presiedere, nel nostro parere abbiamo voluto metterlo bene in evidenza. Abbiamo avuto anche ripetute interlocuzioni con i ministri

avevano una destinazione territoriale specifica, ma molti altri erano a gestione di amministrazioni centrali, quindi con il rischio di perdere una parte delle risorse. In tal senso c'erano stati alcuni allarmi lanciati dagli organi di stampa che lamentavano una perdita di fondi per le Regioni meridionali. Ecco perché sono soddisfatto della previsione contenuta nel decreto-legge, per cui le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR dovranno assicurare il vincolo di destinazione del 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente alle Regioni del Mezzogiorno bandi che prevedano, però, delle clausole, come bene si è impegnata la ministra Carfagna anche in quest'Aula rispondendo a una mia interrogazione. Si tratta di una specificazione doverosa che permetterà a tutte le amministrazioni di operare al meglio per la riduzione di quei divari territoriali che l'Europa ci chiede da troppo tempo di rimuovere, di sanare. Non è conforme ad essa, ad esempio, prevedere un punteggio maggiorato per gli enti che possono offrire un cofinanziamento alle risorse del PNRR. Questo significherebbe infatti che i Comuni del Mezzogiorno sarebbero in parte tagliati fuori dai bandi, visto che sono in situazioni di dissesto e pre-dissesto, e non per responsabilità degli amministratori locali, o almeno non sempre. I divari, così, anziché diminuire, rischiano di aumentare, anzi, aumenterebbero sicuramente. La norma di legge contenuta nel decreto-legge che oggi discutiamo eliminerà questo rischio perché i bandi dovranno vincolare il 40 per cento delle risorse disponibili alle Regioni del Mezzogiorno. Si tratta di una precisazione importante e decisiva che abbiamo molto apprezzato. Il secondo punto su cui mi soffermo velocemente

e spesso suggerendo proposte e temi che io credo abbiano di molto modificato l'impianto che poi abbiamo inviato a Bruxelles e che Bruxelles ha apprezzato. Ora dobbiamo cambiare schema e porci nella condizione di chi dovrà garantire l'effettiva realizzazione dei tanti progetti e delle tante riforme che il PNRR ci assegna come Paese. Le norme approvate alla Camera sul monitoraggio da parte del Parlamento, che forse - lo dico con grande onestà intellettuale - avremmo voluto anche un po' più incisive e che forse dovremo immaginare di completare in corso d'opera, dovranno servire a far sì che tra soggetti attuatori, Governo e Camere si sviluppi una dialettica proficua, nel generale interesse del Paese al completamento dei progetti concordati con le istituzioni europee e all'ottenimento delle relative risorse. L'attuazione del PNRR è una sfida per tutti noi e dovremo essere pronti, anche come Parlamento, a continuare a dare il nostro contributo. È una sfida che non possiamo fallire. Non possiamo fallire nella riduzione delle differenze di genere, generazionali e territoriali. È una sfida

che noi viviamo in quel territorio. Dobbiamo affrontarla insieme, perché i diritti universali e le infrastrutture non sono un tema nelle mani e nelle prerogative degli amministratori locali,

ci aiutino a coltivare la speranza di poter raggiungere un piccolo sogno e di conquistare qualche spazio di civiltà anche nel Mezzogiorno d'Italia.

cittadini, è con profonda amarezza che intervengo sulla conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, constatando che su un provvedimento così strategico per il Paese la centralità del Parlamento è stata nuovamente calpestata. di legge è stato assegnato ieri alle Commissioni del Senato e oggi arriva in Assemblea; nessuna possibilità di presentare emendamenti in Commissione in sede referente, nessuna discussione, neanche il tempo di poter leggere il testo approvato dalla Camera dei deputati. Questo decreto-legge sembra, da una parte, una palese dichiarazione di guerra all'ambiente e, dall'altra, un regalo ai lobbisti e ai criminali ambientali, cui arriva il messaggio che del nostro territorio possono fare quello che vogliono, senza limiti e senza controlli e con i migliori omaggi del Governo Draghi. Questo provvedimento smantella gran parte del minuzioso lavoro svolto per la protezione dell'ambiente e per la salute dei cittadini e mina irreversibilmente i principi che mi hanno sempre guidata nel mio lavoro e nell'esercizio della carica di Presidente della Commissione ambiente. Non potrei, con il tempo che ho a disposizione, elencare tutte le norme scellerate contenute in questo provvedimento, ma almeno alcune di esse devo spiegarle, non tanto a voi che vi apprestate a breve a votare favorevolmente, quanto ai cittadini, che devono sapere chi sono i responsabili dei disastri che da qui a minimo trent'anni si verificheranno. Vi suggerirei, pertanto, di avere la decenza di non fare dichiarazioni di solidarietà nei confronti del popolo sardo, emiliano, campano e di tutte quelle popolazioni che devono subire i danni dei disastri ambientali, naturali e criminali. allora di approfondire qualche articolo. Per effetto delle abrogazioni previste all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, punto 2, viene cancellato il principio secondo cui l'individuazione delle aree per la realizzazione delle opere, degli impianti e delle infrastrutture previste nel PNRR e nel PNIEC deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria, dei corpi idrici e del suolo. Quindi mi chiedo e vi chiedo: come si può parlare di transizione ecologica e di futuro sostenibile del Paese se, pur di realizzare opere e impianti che possono avere impatti ambientali pesanti, lo si fa senza tener conto di criteri così importanti? Semplificare non significa vanificare gli sforzi profusi dagli enti di controllo deputati alle procedure di verifica e valutazione degli impatti ambientali. Anche su questo tema evidenzio che, con l'articolo 19, si invertono i ruoli tra autorità di controllo e proponente, mettendo in capo a quest'ultimo la possibilità di indicare le condizioni ambientali sulle quali l'autorità di controllo si deve esprimere, al fine di non assoggettare un progetto al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Questo significa consentire a chi ha l'interesse economico alla realizzazione dell'opera di proporre all'autorità competente le condizioni ambientali *ad hoc* per poter sfuggire ad una valutazione ambientale più ampia e approfondita. Inoltre, all'articolo 21 è prevista la riduzione dei tempi per la consultazione pubblica da sessanta a trenta giorni, mortificando di fatto i cittadini e impedendo loro di partecipare per poter decidere sulle sorti del proprio territorio. La consultazione pubblica è un principio mutuato dalla direttiva UE n. 52 del 2014 in materia di VIA e rappresenta uno strumento fondamentale per garantire un confronto moderno, democratico e trasparente. Togliamo un diritto ai cittadini, da una parte, e facciamo un bel regalo ai lobbisti, dall'altra. Lo stesso avviene per il fotovoltaico, all'articolo 31. La norma vigente prima del decreto prevedeva che la realizzazione di impianti fotovoltaici in aree industriali non fosse sottoposta alla verifica di assoggettabilità a VIA per impianti fino a un questo limite è stato portato a 10 megawatt e addirittura innalzato a 20 megawatt alla Camera. Questi megaimpianti, che potranno tra l'altro essere realizzati anche in discariche o cave dismesse, non possono non avere ricadute irreversibili sul paesaggio e l'ambiente. l'ambiente. Ma voi avete tolto anche la possibilità di verificarlo, impedendo qualsiasi progetto di recupero ambientale. All'articolo 33 avete macchiato una norma buona come il superbonus 110 concedendo ai proprietari di immobili parzialmente o totalmente abusivi di ricevere gli incentivi, inventandovi una "bella" sanatoria generalizzata. Ovviamente, quegli edifici che stavano per essere demoliti perché abusivi ora resteranno dove sono, perché lo Stato gli dà pure gli incentivi: ottimo messaggio per gli abusivi, complimenti. Gli ultimi due articoli, a cui tengo maggiormente perché sono i peggiori di tutti, sono il 34 e il 35. All'articolo 34 si parla di *end of waste* e non potete non ricordarvi quanto siamo riusciti, dopo tanto lavoro, ad approvare durante il Governo Conte II: una norma che aggiungeva al testo unico ambientale l'articolo 184-*ter*; una norma che aveva sbloccato uno stallo cronico e riformato la normativa sull'*end prevedendo che le autorizzazioni per i processi industriali che portano alla cessazione della qualifica di rifiuto potessero essere rilasciate caso per caso dalle Regioni e dalle Province, che si dovevano però attenere a quanto previsto dalla direttiva europea di riferimento (la direttiva CE e ai requisiti che avevamo inserito nella norma stessa. Ma avevamo anche previsto un sistema di monitoraggio e di controllo da parte dell'ISPRA e delle ARPA regionali che, a campione e *post* autorizzazione, avrebbero dovuto verificare che negli impianti semplicemente avvenisse ciò per cui erano stati autorizzati, pena il ritiro dell'autorizzazione se non fossero stati in regola. L'articolo 34 del decreto-legge semplificazioni cancella di fatto i commi dell'articolo 184-*ter* in tema di controlli. Mi chiedo: se questo decreto è stato voluto soprattutto per semplificare e accelerare le procedure delle autorizzazioni, perché cancellare i controlli che invece sono previsti dopo aver avuto l'autorizzazione? Probabilmente chi deve operare nella miscelazione dei rifiuti non voleva essere disturbato e voi lo avete accontentato. Pensate alla responsabilità dei danni alla salute che ne deriveranno e che vi siete assunti. In ultimo, mi soffermo sull'articolo 35 contenente misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare. I commi 2 e 3 non sono altro che un enorme e ingiustificato regalo alle *lobby* delle cementerie. Consentire la sostituzione dei combustibili tradizionali con combustibile solido secondario (CSS), che altro non è che rifiuto, in impianti o installazioni già autorizzati, senza che ciò rappresenti una modifica o una variante sostanziale dell'autorizzazione, rappresenta un serio pericolo e un affronto ai tanti, tantissimi cittadini e comitati che in questi anni si sono rivolti alle istituzioni con una disperata richiesta di aiuto. Grazie al famigerato decreto Clini, nel 2013, il CSS è diventato magicamente un *end of waste*. Si è permesso che questi rifiuti venissero bruciati nei cementifici, ma questi sono impianti che, a livello tecnico, non sono dotati di idonei sistemi di abbattimento degli inquinanti contenuti nei fumi e quindi sono addirittura più pericolosi degli inceneritori. Il paradosso ancora più grande è però che la direttiva europea n. 851 del 2018, relativa ai rifiuti, stabilisce che i rifiuti utilizzati come combustibile non sono computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. Quindi, a quale norma di promozione dell'economia circolare si riferisce questo articolo 35? Queste sono solo alcune delle misure nefaste contenute in questo decreto-legge. Ora veniamo al commento politico. Alle altre forze politiche non mi rivolgo, perché da sempre sognavano un decreto di tale portata, ma ai miei ex colleghi del MoVimento 5 Stelle sì. Ricordate nel novembre 2014? Votammo il decreto cosiddetto sblocca Italia di Renzi, nel quale, fra le varie cose, si dichiaravano strategici inceneritori e trivelle. Noi ci opponemmo e per questo molti di noi furono puniti con la sospensione dei lavori di Aula e Commissione per dieci giorni e fummo anche denunciati alla procura della Repubblica per aver rallentato il voto in Aula. Lo sblocca Italia non è niente in confronto a quello che è previsto in questo decreto-legge. Mi chiedo allora come sia possibile che rimaniate in ossequioso silenzio e siate pronti a votare favorevolmente questo decreto che annienta quella che era la nostra prima stella, l'ambiente. La coerenza nei principi e la salvaguardia dell'ambiente era ciò che ci contraddistingueva da tutto il resto. Voi vi siete piegati e vi siete assuefatti al sistema; avete venduto la stella dell'ambiente alla bancarella di Draghi in cambio di che cosa? Questo è un tradimento che gli italiani non vi perdoneranno e di certo neanche io. rappresentante del Governo, colleghi, oggi siamo in quest'Aula per approvare e rendere operativo un decreto che nel suo titolo un decreto che nel suo titolo informale contiene una parola d'ordine, un imperativo categorico, un termine che farà la differenza tra lo sviluppo e la crescita del Paese rispetto alla possibilità nefasta di rimanere al palo. Questa parola è «semplificazione», la prima grande riforma senza la quale perdono senso tutte le altre. Nella tragedia sanitaria, nella difficoltà sociale ed economica del Covid, un effetto un effetto positivo la pandemia lo ha prodotto: si è ingenerata finalmente la consapevolezza dello stato di necessità del Paese rispetto a un sistema burocratico ormai diventato un'armatura di gesso, ingestibile, paralizzante. L'Italia è il Paese che ha fatto dell'ingegno la propria materia prima. È un Paese la cui ossatura è formata dalle piccole e medie industrie, dal manifatturiero, dalle attività produttive. È un Paese in cui la libera iniziativa produce capolavori, ma è anche un Paese dove la capacità di creare prodotto e lavoro viene frenata, messa in difficoltà osteggiata da un sistema burocratico complesso, ingiustificato e ormai pletorico per un Paese che non solo deve dimostrare resilienza - termine che vuol dire tornare come si era - ma necessita di crescere e di evolversi. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza - lo abbiamo sostenuto, ripetuto e continueremo a ripeterlo - è un'occasione unica per rilanciare il Paese, che dovrà dimostrare di saper trasformare un debito in *leverage*, in una leva per produrre redditività, crescita e lavoro. È stato molto chiaro il presidente Draghi nel suo discorso di insediamento, nel suo passaggio darwiniano. Il Governo sosterrà l'intraprendenza, cioè chi saprà dimostrare non solo di resistere passivamente, come dicevo prima, di tornare come prima, ma di sapersi evolvere. Il provvedimento oggi esame necessiterà di ulteriori passaggi e altri momenti. Questo è un primo *step*. Il Senato oggi non ha la possibilità di esprimersi come vorrebbe e questo ormai è un dato di fatto; allo stesso tempo domani dovremo esaminare un altro provvedimento importante, che è quello sul reclutamento, dove abbiamo abbiamo avuto noi la possibilità di intervenire. Quindi, ognuno fa la propria parte in questo sistema integrato. Questo provvedimento è comunque la fionda che aspettavamo per consentire di scardinare l'armatura soffocante che opprime il Paese, che impedisce ai tanti ingegnosi di realizzare gli obiettivi di crescita e creare nuovi posti di lavoro. Per far marciare rapidamente il PNRR era indispensabile eliminare i colli di bottiglia che avrebbero potuto ritardare gli investimenti, l'attuazione dei progetti, mettendo a rischio l'intera strategia per il rilancio del Paese o almeno cominciare a farlo. Grazie a questo provvedimento, che è la prima pietra miliare del PNRR, l'Italia potrà ottenere a breve l'anticipo di 25 miliardi sui circa 200 miliardi di fondi UE che spettano al nostro Paese.

L'opposizione dice che ci sono tanti articoli: ebbene, ci sono tanti articoli perché ci sono tante semplificazioni, tanti temi, tanti argomenti che meritavano di essere di essere toccati e semplificati. È evidente quanto questo decreto sia decisivo per realizzare le opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche per determinare un cambio culturale e strutturale del nostro sistema statale, fattore decisivo di competitività, visto che da diverse analisi, in particolare quella dell'ufficio studi di Confcommercio, le inefficienze della pubblica amministrazione incidono in modo diretto sulla crescita dell'economia nazionale, con una perdita di circa 70 miliardi di PIL. Questo non ce lo possiamo permettere. Il *recovery plan* è forse la più grande sfida di modernizzazione che il nostro Paese si trova ad affrontare dal dopoguerra, una sfida di grande ricostruzione dopo una lunga crisi aggravata da questa terribile pandemia. Quindi, noi oggi, pur dispiaciuti di non aver potuto dare un ulteriore contributo, ma sicuramente consapevoli che non mancheranno future occasioni, siamo contenti contenti che la semplificazione non sia più soltanto una parola, ma diventi effettivamente e oggettivamente un percorso e una realtà.

che cosa avessero intenzione di fare: se essere un filtro tra il privato e il risultato da raggiungere, oppure se essere uno strumento tra il progetto da realizzare e il privato cittadino. un po' una provocazione, un po' un ragionamento filosofico, che però aveva delle implicazioni profonde, perché è evidente a tutti che se la pubblica amministrazione inizia a collaborare con il privato nel perseguimento del proprio obiettivo, obiettivo, la realizzazione avviene in tempi più rapidi e in maniera più efficace. Finalmente, dopo venti anni, ecco un provvedimento che va nella direzione da me auspicata: finalmente, perché si punta a cambiare punta a cambiare quello che sarà il rapporto tra pubblica amministrazione e privati, perché è quello che serve al Paese. Sappiamo tutti che questo provvedimento è funzionale al PNRR. Sappiamo tutti che le risorse del *recovery plan* dovranno essere spese entro il 2026, ma sappiamo tutti altrettanto bene che l'Italia non è mai stata brava a spendere rapidamente e bene le risorse o quantomeno non lo è stata fino a che la Lega non è diventata motore trainante di un Governo. *(Applausi)*. del ponte Morandi, reduci dall'esperienza del terremoto del Centro-Italia del 2016, quella che all'epoca definivo come la base di una delle peggiori ricostruzioni d'Italia; i fatti poi mi hanno dato ragione, visto che a cinque anni stiamo iniziando ora a ripartire, anche grazie alle semplificazioni che sono state introdotte nel frattempo. Come dicevo, ciò è avvenuto finché la Lega non ha deciso di cambiare il paradigma e introdurre un modello

indicato da tutti come modello di efficacia ed efficienza non solo per la ricostruzione di un ponte, ma anche per ciò che diventerà il nostro vero *recovery plan,* il nostro vero decreto ristori. Infatti, la possibilità di spendere in maniera rapida ed efficace le risorse del *recovery plan* ci consentirà di creare centinaia di migliaia di posti di lavoro.

e potrò permettermi solo di accennare ad alcune di esse, rispondendo anche a coloro che vedono sempre il bicchiere mezzo vuoto. A mio avviso, è un problema in parte anche caratteriale, di cultura politica e personale e non tanto perché la Lega non veda il bicchiere mezzo vuoto. Anzi, io personalmente, ma anche la Lega vediamo sempre il bicchiere mezzo vuoto ma non già per puntare il dito e criticare, bensì per cercare di migliorare i provvedimenti e fare quello che serve e che anche in questo caso è stato fatto grazie alla collaborazione dei colleghi della Camera Non sto dicendo che il provvedimento è perfetto e realizza tutto quello che avremmo voluto (personalmente, nemmeno sarei capace di realizzare un provvedimento perfetto).

è certo che questo provvedimento è utile. Anzi, vado oltre dicendo che questo provvedimento per me è indispensabile perché introduce misure in un settore

voglio iniziare il mio discorso riportando la vostra attenzione sul *summit* G20 che si è tenuto a Napoli, che ha visto protagonisti i Ministri dell'ambiente e dell'energia dei Paesi più ricchi del mondo. La conferenza aveva come scopo quello di rilanciare e rafforzare gli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi del 2015, soprattutto in vista del vertice delle Nazioni Unite sul clima, la COP26. Molti hanno detto che l'accordo è stato un fallimento, ma non è così. È giusto ribadire che lo *staff* del Ministero della transizione ecologica e lo stesso ministro Cingolani sono riusciti a portare a casa 58 punti all'ordine del giorno su 60 e questo è un è un grande successo per l'Italia; come ha detto in un'intervista il Ministro, aver convinto i grandi ad affrontare insieme quei temi è stata una novità assoluta, da considerare come un successo della Presidenza italiana, come d'altra parte ci è stato riconosciuto da tutte le delegazioni. Certo, c'è da dire che non è un successo per quelle Nazioni che, come al solito, si sono svincolate; l'hanno fatto anche nei *summit* mondiali gli altri anni, nelle altre COP - lo ricordo bene, quando ho partecipato con il ministro Sergio Costa alle ultime due - mentre l'Italia, anche allora, è stata sempre esemplare sui trattati internazionali. Tutti i Paesi hanno concordato che, soprattutto dopo la fase pandemica, la transizione energetica verso le energie rinnovabili è uno strumento per la crescita socio-economica, inclusiva e veloce, per la creazione di posti di lavoro. È una transizione giusta che non lascia nessuno indietro. La comunità internazionale del G20 riconosce nella scienza un ruolo fondamentale su cui la politica deve basarsi e soprattutto viene riconosciuto uno stretto nesso tra clima ed energia e la necessità di ridurre le emissioni globali e migliorare l'adattamento al cambiamento climatico, quello che sta causando tutto quello che stiamo vedendo in Italia e anche in altri Paesi in questi giorni. Rimane centrale il ruolo dell'impegno finanziario dei 100 miliardi, così come previsto dall'Accordo di Parigi, con l'impegno di aumentare i contributi ogni anno fino al 2025. La transizione, quella vera, è necessaria e indispensabile, ma dev'essere appunto giusta e assicurare sostegno e solidarietà alle categorie e ai Paesi più fragili. Vi ho parlato di questo perché è chiaramente collegato a quello che oggi stiamo dicendo in Aula, dove stiamo parlando del decreto semplificazioni, che ovviamente è collegato all'obiettivo di neutralità climatica. climatica. Lasciatemi prima di tutto ringraziare tutti i colleghi e le colleghe della Commissione ambiente della Camera, che hanno lavorato duramente in queste settimane su questo importante provvedimento. Il MoVimento 5 Stelle è stato impegnato costantemente per introdurre norme più coerenti con la transizione ecologica rispetto alla prima stesura del testo

ma qui non ho trovato semplificazioni per controllare e supportare le decine di nuovi prodotti che richiedono nuove tecnologie per poter procedere al loro riciclo. Non ci sono semplificazioni per migliorare le percentuali di raccolta differenziata e di riciclo; mi aspettavo qualcosa anche sulla simbiosi industriale, ma non c'è. Nell'Allegato I-*bis*, invece, nell'elenco delle opere strategiche per il Piano nazionale integrato energia e clima 2030, inseriamo nuovi impianti per la produzione di energia da residui e rifiuti. Vi dico che non servono.

dobbiamo essere noi a gestirlo. Dagli ultimi rapporti ISPRA sulla gestione dei rifiuti, però, l'Italia è al *top* europeo per riciclo e recupero di materia e, di conseguenza, c'è stata una riduzione del numero di impianti che bruciano rifiuti dell'11 La tecnologia, la raccolta differenziata e la collaborazione dei cittadini stanno riducendo la necessità di incenerire i rifiuti, allora perché costruirli?

parliamo di decarbonizzare e poi vogliamo aprire nuovi inceneritori? Tutto ciò non è coerente. Non c'è coerenza neanche con le priorità stabilite dalla Commissione europea per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con il principio *do no significant harm* (non arrecare alcun danno significativo). Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo lavorato nel processo emendativo per migliorare il testo e siamo riusciti a vincere alcune battaglie: dai vaccini all'ambiente, dal superbonus ai risparmi in bolletta per i cittadini. C'è la norma che regola e frena l'eolico selvaggio, quella che consente di fissare piccoli impianti fotovoltaici anche su strutture diverse dagli edifici. Penso altresì all'emendamento sul deposito cauzionale per regolarizzare e migliorare il recupero degli imballaggi, per continuare dunque la nostra battaglia *plastic free,* per recuperare vetro e alluminio come richiesto richiesto dagli obiettivi del decreto legislativo n. 116 del 2020 sull'economia circolare. Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza con un nostro emendamento garantiamo un maggior controllo sulla gestione dei fondi del *recovery plan,* valorizzando il ruolo dell'Autorità nazionale anticorruzione. Le famiglie non si ritroveranno più in bolletta oneri che derivano da debiti non pagati da alcuni venditori e che finora venivano coperti smaltendoli su tutti i cittadini: milioni di euro finora caricati sui cosiddetti oneri generali del sistema ora diventeranno risparmio per le famiglie. Il MoVimento 5 Stelle ha dimostrato anche in questa occasione di essere una forza politica responsabile e attenta ai bisogni dei cittadini e dell'ambiente. Continuiamo a svolgere il nostro compito di custodi dei nostri territori e a essere un'unica comunità che deve andare oltre la crisi e guardare con speranza e serenità al 2050. Il MoVimento 5 Stelle c'è e ci sarà sempre. Dichiaro chiusa la discussione generale. Il rappresentante del Governo non intende intervenire Signora Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico

La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 77, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito. Sospendo

una nuova finestra"). La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante *governance* del PNRR e semplificazioni, nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, che avranno luogo domattina alle ore 9,30. Seguirà la chiama. Dopo la chiama la seduta sarà sospesa per riprendere alle ore 16,30 con la discussione del decreto-legge sul rafforzamento delle pubbliche amministrazioni e della giustizia. Giovedì 29 luglio, alle ore 15, si terrà il *question time*, con la presenza dei Ministri degli affari esteri, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute. Nella settimana dal 3 al 5 agosto saranno discussi i decreti-legge sulla cybersicurezza, attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati, e sulla salvaguardia di Venezia. Il calendario prevede inoltre le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126*-bis*, comma 2*-bis*, del Regolamento, sul disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica concernente delega al Governo in materia di spettacolo, nonché la discussione dei disegni di legge rendiconto 2020 e assestamento 2021. Giovedì 5 agosto alle ore 15 si terrà il *question time.* Il calendario della prossima settimana potrà essere integrato con la discussione di atti di indirizzo concernenti la partecipazione dell'Italia a missioni internazionali,

Grazie